sostegno.

Prego,

ed il licenziamento delle maestranze. E[]un argomento rilevante e significativo. Per una ragione di coerenza rispetto agli impegni che ieri il Governo ha assunto di fronte

Qui fissiamo un tasso di inflazione all’1,7 per cento quando sappiamo che il tasso di inflazione reale esuperiore. con questo emendamento e cercare di sensibilizzare anche i colleghi della maggioranza perche´ non puo essere fissato un tasso di inflazione per i lavoratori dipendenti, anche quelli del pubblico impiego, all’1,7 per cento.

In questo caso ritireremmo l’emendamento.

Presidente, l’emendamento 2.345 affronta il problema molto serio, che abbiamo sollevato in Commissione chiedendo al Governo dati e una presa di posizione piuprecisa, che e la nota questione dell’integrale ristoro dell’ICI ai Comuni. Ne abbiamo discusso piuvolte in Commissione, piu volte in Aula, il Governo si eimpegnato a restituire integralmente queste risorse ai Comuni, lo ha fatto con l’approvazione del decreto sull’ICI, accogliendo peraltro, in quella circostanza, un ordine del giorno, lo ha fatto in occasione dell’approvazione del decreto-legge n. 112, da ultimo con il decreto-legge decreto nel quale era recato lo stanziamento di 260 milioni di euro, che costituiva pacificamente un acconto ulteriore I Comuni italiani, com’e noto, sono in rivolta, l’ANCI ha invitato i Comuni a non approvare i bilanci entro il termine di legge fissato al 31 dicembre, fino a quando il Governo, appunto,

moltissimi Comuni rischiano di non poter chiudere i bilanci, di non poter approvare i bilanci previsionali del 2009 in equilibrio e quindi con rischio di dissesto finanziario, di decurtazione dei servizi; il tasso di federalismo, com’enoto, praticamente compromesso, quindi si tratta di un vero e proprio capolavoro sulle politiche di bilancio e di finanza pubblica che richiederebbe un chiarimento urgente. Peraltro, essendo pacifico che i Comuni avranno diritto, allorquando ci sara` la certificazione definitiva delle minori entrate, all’integrale restituzione, si rischia anche di creare un buco nel bilancio dello Stato. So che il Governo ha intenzione di farlo, il sottosegretario Vegas ce lo ha detto in Commissione, ma questa misura, come da impegno, doveva essere adottata entro il 31 dicembre.

Questo ovviamente non deve valere da pretesto per non approvare i bilanci o per non adempiere al Patto di stabilita, perche´ ovviamente sarebbe un fuor d’opera rispetto a questo lavoro che stiamo facendo per salvaguardare gli interessi di tutti. poiche´ il Governo ha ribadito in Aula questo impegno, credo che non avradifficolta ad accogliere un ordine del giorno in tal senso, in maniera che si sappia il Governo eimpegnato, entro tempi ragionevoli, a soddisfare questa legittima richiesta dei Comuni italiani. Chiedo quindi la disponibilita ad accogliere un ordine del giorno in tal senso.

perche´ il Governo si impegni, in un prossimo provvedimento destinato agli enti locali, a prendere in considerazione questo tema delicatissimo della sicurezza delle scuole, che puo essere assolto dagli enti locali qualora vengano messi nelle condizioni di poter spendere le risorse a loro disposizione che, per ora, non possono utilizzare perche´ vincolati dal Patto di stabilita. Per quelle somme che come avanzi di amministrazione possono essere utilizzate come investimenti per la sicurezza delle scuole credo che il Governo possa accettare un ordine del giorno per un prossimo provvedimento e per il prossimo Patto di stabilita.

a questa falcidie dei nostri emendamenti. Ma su questo in particolare vorrei richiamare l’attenzione del Governo. La scorsa settimana, quando quest’Aula ha licenziato il decreto-legge sulla competitivitanel settore agroalimentare, dopo alterne vicende in contraddittorio tra la Presidenza, il relatore ed il rappresentante del Governo quanto alla copertura finanziaria del Fondo di solidarieta nazionale per il solo anno 2008 (copertura che poi estata fissata in

del Senato avesse licenziato un provvedimento con la relativa assicurazione della copertura finanziaria e che poi diversamente venisse disposto alla Camera dei deputati. Cio significherebbe

del quale ho una grandissima stima anche per la sua consueta correttezza, che il Governo sta dimostrando la massima attenzione nei confronti dei problemi dell’agricoltura. Ciosi puo evincere da una serie di iniziative intraprese sia a livello nazionale che a livello comunitario. I successi del ministro Zaia, propiziati anche dall’intervento del presidente Berlusconi, per quanto riguarda la partita delle quote latte, sono dinanzi a tutti noi.

Presidente, stanti le assicurazioni ricevute dal ministro per la semplificazione legislativa, senatore Calderoli, data l’improprieta della sede, per cui il Governo ha espresso parere contrario su questo emendamento, lo ritiro,

Presidente, faccio una breve dichiarazione di voto perche´ l’argomento edi rilievo e so che anche colleghi della maggioranza si sono posti il problema, sia alla Camera che qui al Senato, della cooperazione internazionale. internazionale. Con questa scelta la cooperazione internazionale scende nei programmi del Ministero degli affari esteri (e non dovrebbe essere l’opposizione a difendere i programmi del Ministero degli affari esteri)

Allora, chiedo con questo emendamento un aumento di soli 9 centesimi su questo pacchetto di sigari (e io sono un fumatore).

restituire almeno 200 milioni alla cooperazione. Questa e la scelta che chiediamo a tutti. Non cito i colleghi della maggioranza perche´ capisco la loro situazione, ma ritengo sia giusto che cio` si sappia. (Applausi

Fondo diventato oggetto di tanti commenti politici, di tante riflessioni parlamentari,

con una elencazione puntuale di tutte le risorse che sono state, se non sottratte, quanto meno prelevate dal FAS ed utilizzate per le piusvariate attivita.

Il fantasma piu disastroso dell’economia meridionale erappresentato dalle Ferrovie dello Stato, con la loro assenza cronica, con il loro disimpegno perfino sulla qualita dei servizi, che sono

problemi di particolarissima delicatezza con riferimento alla significativita del bilancio a legislazione vigente, cosıcome lo stiamo discutendo e approvando.

l’utilizzo del FAS per finalita improprie, che giasi e determinato sulla base della legislazione vigente,

e ammonta al 50 per cento delle risorse disponibili. Signor Presidente, richiamo anche la sua attenzione perche´ si tratta di un problema che riguarda i nostri poteri e la significativita della decisione dell’Assemblea sul bilancio di previsione a legislazione vigente. Secondo questa nota della Ragioneria, le disponibilitafissate in bilancio per il 2009 a proposito del FAS ammontano, per la precisione, a 5.999.110.000 euro. Segue, nella nota della Ragioneria che adesso per brevita non leggo, la elencazione puntuale, come da nostra richiesta in Commissione bilancio, degli utilizzi del FAS per finalitaimproprie. Il risultato

cioecirca 6 miliardi di euro; in realta, la Ragioneria generale dello Stato documenta alla Commissione bilancio che le risorse ammontano a meno di 3 miliardi di euro: questa euna situazione nella quale si pone un serio problema, che riguarda la significativita e il rilievo della decisione parlamentare su una delle componenti fondamentali della spesa in conto capitale del bilancio della Repubblica.

il federalismo nel Paese, compiamo un atto che eesattamente opposto a quello che il Governo, il Parlamento e gli amici della Lega vogliono fare.

Signor Presidente, vorrei ricordare alla Presidenza e all’Assemblea che l’intero Gruppo del Popolo della Liberta, estremamente preoccupato per l’andamento dell’utilizzo del fondo FAS, dicembre 2008 una mozione perche´ si attivi una discussione ad hoc in Aula sull’argomento e perche´ il Governo indichi quali sono i provvedimenti con i quali intende ripristinare l’intera dotazione del fondo FAS che interessa, come

Non mi sembra tuttavia, pur essendo d’accordo sulle considerazioni di fondo e di merito svolte dai senatori Pistorio e Cuffaro, che il meccanismo di questo emendamento risolva il problema. Quindi, in questa sede il Popolo della Libertanon votera

Penso che abbiamo giaillustrato sufficientemente questi tre emendamenti gia nella giornata di ieri, anche in quell’occasione con una sola presentazione. Sarebbe utile che il Governo facesse una riflessione veloce su uno dei tre, anche via anche via sms, purche´ la riflessione porti ad un risultato positivo. Ricordo al relatore e ai rappresentanti del Governo che il primo di questi emendamenti euna richiesta one shot, come si usa in gergo, di esporre per l’Abruzzo, utilizzando i fondi FAS, interventi solo per il 2009 sulla ferrovia e sui bacini idrici del Fucino, fermi da circa trent’anni. Il secondo emendamento e piuimpegnativo perche´ e una richiesta di intervento per tre anni con un fondo di 200 milioni di euro. Il terzo ripristina cioche il Governo Berlusconi ha tagliato nella prima occasione in cui poteva farlo, cioe distogliendo

e ben strano che il nostro Presidente del Consiglio – ho usato volutamente la parola «nostro» che mi estata da qualcuno rimproverata nella notte passata, ma ritengo che il Presidente del Consiglio, ancorche´ eletto da una parte del Parlamento e il Presidente del Consiglio degli italiani

per gli affari regionali, ad innumerevoli rappresentanti importanti e quotati del Governo, a dire la stessa parola: bisogna investire in infrastrutture in quella Regione.

se vuole le dico subito che il meno costoso eil 2.411, il piu impegnativo in termini di infrastrutture ma il meno costoso in termini di oneri – penso farebbe un’ottima figura nei confronti dei cittadini abruzzesi. Ci interesserebbe sapere se il Governo e` disposto a cambiare idea su uno di questi tre emendamenti.

in vista del voto regionale di domenica prossima, perche´ sappiamo benissimo che i fondi, ove concessi in assenza di una progettualita e di una documentazione

la dotazione che era stata prevista per la tratta ferroviaria Avezzano-Roma e che poi, nella realta, si riscontronon essere utilizzabile proprio perche´ non esisteva alcun progetto per l’ammodernamento di quel collegamento.

un intervento infrastrutturale per tutto il sistema Paese, e proprio l’Abruzzo che rappresenta la cerniera tra Nord e Sud e tra Est ed Ovest della nostra penisola. Quindi, l’impegno c’e. Pertanto,

queste problematiche in modo serio e mi auguro che in quella sede l’opposizione ci dia anche una mano.

questo Governo ha tagliato i fondi per collegamenti giastanziati e gia finanziati. Lo ripeto ancora una volta,

ma anche gli altri, sappiano che le promesse sono una cosa e i fatti sono altra cosa. Per tale ragione, oltre a sottoscrivere questi emendamenti,

quindi con raccomandazioni e con conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti. Nel frattempo, il fondo FAS viene tagliato e utilizzato in modo improprio. Con questo emendamento, comunque, affrontiamo un altro tema sempre legato al fondo FAS, cioe la capacitadi spesa reale che bisogna comunque dimostrare e quindi anche l’incidenza che il fondo FAS realmente deve avere sui territori e in modo particolare sul Mezzogiorno. Con questo emendamento proponiamo una soluzione. Ci sono dei fondi FAS che sono nelle mani delle amministrazioni centrali, sottolineo centrali, che non sono stati utilizzati.

di un emendamento che penso potrebbe essere accolto ed e ben strano che anche su questa metodologia selettiva e innovativa ci sia un netto rifiuto da parte del Governo.

con altri 110 Paesi. Tuttavia, sarebbe incoerente impegnarsi in un trattato importantissimo e contestualmente togliere i fondi sullo sminamento.

e che occorre fare opera di prevenzione per contenerla e opera di accoglienza delle donne vittime della violenza, spesso donne con bambini. L’accoglienza viene svolta dai centri antiviolenza,

che incidentalmente e anche il possessore della comunicazione televisiva privata e il controllore di quella pubblica, prende provvedimenti per tagliare i fondi all’editoria. invece, che vengano salvaguardati i fondi per l’editoria. Quale guadagno la democrazia puoricavare dalla chiusura dei piccoli giornali, dalla chiusura dei piccoli giornali, delle piccole attivita editoriali? Si vuole determinare un panorama grigio, uniforme, dove esiste soltanto la grande editoria che non ha bisogno di sostegno.

I colleghi della Lega dovrebbero pensare un po’ al destino della loro stampa, anch’essa in pericolo perche´ non ha la statura di grande impresa. E[` ]un punto fondamentale su cui lo sventurato emendamento

Presidente, intervengo per una duplice ragione: oltre a motivare il mio voto favorevole a questo emendamento, desidero anche porre una questione formale, che ho giaposto ieri su un caso abbastanza simile. Si trattava di alcuni emendamenti relativi al Belice, giudicati inammissibili dalla Commissione perche´ localistici, mentre il testo del Governo, all’articolo 2, comma 9, prevede una norma di contenuto

sul Belice, pur nel massimo rispetto per il presidente della Commissione, l’amico Azzollini. Accade ora la medesima cosa: estato ammesso l’emendamento 2.468 ed e stato giudicato inammissibile il 2.467, il 2.467, che prevedeva una norma ragionevole: per una sperequazione o una discrasia legislativa, i benefıci relativi alla sospensione

infatti, sono incappate nell’errore di considerare sospesa anche la parte contributiva, mentre vi era soltanto la sospensione per quella tributaria. L’emendamento, dunque, prevedeva l’allineamento temporale, mettendo in sintonia due provvedimenti del Governo, un decreto-legge che riguardava la sospensione dei meccanismi contributivi e un decreto ministeriale che riguardava la parte tributaria.

con un’individuazione dei luoghi dove operare a carico del Ministero dell’economia di concerto con il Ministero dell’agricoltura. Questo e un altro di quegli interventi utili e idonei, finanziabili con il Fondo per le aree sottoutilizzate.

che questi siano emendamenti spot, asserendo che indicare delle cifre sia un mero esercizio di stile in assenza di una progettazione. Come se i componenti

non avendo sentito alcun intervento da parte del Governo in materia e siccome continuo a ricordare al rappresentante del Governo, che pure e` impegnato in assidue discussioni, che il suo ed il nostro Presidente del Consiglio va e promette come fanno altri, probabilmente questo Governo dovrebbe cominciare a dare un segnale (anche perche´ andate alle elezioni, senatore Pastore)

vista l’assenza totale di impegni sugli altri argomenti.

l’emendamento 2.520 interviene su un altro tema imbarazzante, rappresentato dalla disponibilitadei fondi per le vittime del dovere e i loro familiari I fondi sono gia scarsi, ma vengono ulteriormente ridotti. Si avverte una stringente contraddizione tra la retorica parlamentare e la prassi: la prima si diffonde in elogi gratis alle Forze dell’ordine, ai soldati all’estero e a tutti coloro che compiono il proprio dovere per salvaguardare l’integritadello Stato; quando pero si tratta di devolvere il minimo delle somme necessarie, la borsa si chiude.

certo): estata in pericolo la disponibilita dei fondi a sostegno delle vittime dell’uranio impoverito. Probabilmente si riusciraa porre rimedio; il Sottosegretario

chiesto il voto elettronico

si tratta di una politica un po’ diversa da quella del Governo, si puo` accogliere come raccomandazione indicativa, ma prendendola molto con le molle.

Ne ha facolta`. PARDI (IdV). L’emendamento chiede, contrariamente all’orientamento della maggioranza e del Governo, che siano aumentati i finanziamenti a vantaggio dell’universitae della ricerca, perche´ si ritiene che la possibilita di uscire in modo significativo dalla crisi economica dipenda assai piudall’investimento nella conoscenza e nella ricerca scientifica piuttosto che in attivita dispersive e di scarsa fortuna.

Il Senato non approva.

Poiche´ tale incongruenza puo essere risolta anche in sede interministeriale, sono disposto a ritirare i due

una totale sorditada parte del Governo. Avevamo rilevato – e ci sono indagini ulteriori in questi giorni che lo confermano – un momento di grave sofferenza nel comparto agricoltura e pesca e pensavamo di poter dare un sostegno e un supporto utili per il loro rilancio anche in questa circostanza, dopo il tentativo fatto in sede di approvazione

relativo alla viabilita non statale nelle Regioni Sicilia e Calabria che fu oggetto di un confronto serrato con il Governo del tempo, quello presieduto dall’onorevole Prodi, e che vide in grande sintonia le amministrazioni locali – le Regioni, le Province e i Comuni di Sicilia e Calabria – nella volontadi rendere concreta una norma della legge finanziaria che il Governo Prodi aveva varato, ma che poi era stata disattesa, come altre, dal Ministero dell’economia. Allora attorno a questo finanziamento si scateno – possiamo dire cosı– una battaglia bipartisan che riguardo le due Regioni e le loro amministrazioni e che ebbe il suo momento piuvigoroso in una manifestazione pubblica davanti a Palazzo Chigi, con la mobilitazione di qualche migliaio di cittadini calabresi e siciliani che giunsero a Roma per chiedere che quel finanziamento fosse attivato. A margine di quella

nostro Governo, con uno dei suoi primissimi provvedimenti, quello relativo alla copertura dell’ICI, ha ha revocato quei finanziamenti, lasciando in notevole difficolta le amministrazioni che, dovendo beneficiare di un finanziamento triennale, avevano giaprogrammato le risorse per le opere nel triennio.

distratte con urgenza per finanziare la copertura dell’ICI su tutto il territorio nazionale sarebbero state riattribuite alle Regioni Sicilia e Calabria. Vorrei che il Governo avesse un ripensamento onesto, visto che in tutte le sedi c’estato garantito questo provvedimento, e cogliesse tale occasione come un’opportunita per chiudere questa partita, francamente imbarazzante.

un problema che, ripeto, sta diventando sempre piu drammatico per il sistema delle autonomie locali. Proprio ieri, il presidente dell’ANCI e il governatore della Banca d’Italia si sono incontrati per stimare,

che consenta, da un lato, di introdurre norme finalizzate ad obbligare alla rinegoziazione di questi strumenti, dall’altro, di vietare totalmente per il futuro la stipula di contratti di questa natura, che comportano rischi molte volte insopportabili per il bilancio degli enti locali.

una chiarificazione su tale materia e consentire quantomeno di accertare qual e il deficit sommerso che si eaccumulato nel corso di questi anni, deficit degli enti locali e delle Regioni che si aggiunge a quello derivante dalla omessa reintegrazione del trasferimento ICI, dalla vicenda ICI sui fabbricati rurali, dalle riduzioni dei trasferimenti operati con il decreto-legge n. 112 e quant’altro. Vi e una situazione veramente difficile per il sistema delle autonomie locali e la questione dei derivati rischia

Detto questo, il Governo e intervenuto appena insediato e con il decreto-legge n. 112 ha emesso una norma di blocco temporaneo; ovviamente non poteva fare diversamente. L’emendamento del relatore, l’attuale articolo 2-bis, consente, da una parte, di tenere fermo il blocco, permettendo nel frattempo la rinegoziazione

il meccanismo che e previsto nell’emendamento presentato dal relatore in Commissione consente, in qualche modo, di salvaguardare il piupossibile la posizione degli enti locali, rendendosi conto che si tratta di un tema molto delicato. comunque, che il Governo eapertissimo a considerare eventuali possibili miglioramenti, sempre nell’ambito della salvaguardia complessiva dei sottoscrittori, soprattutto nel caso in cui la loro buona fede sia stata tradita; tuttavia bisogna tenere presente che nei meccanismi di mercato

se noi controlliamo la prima pagina economica del «Corriere della sera» di oggi, leggiamo il titolo: «Caos derivati per i Comuni», vertice tra il governatore della Banca d’Italia e il presidente dell’ANCI. Ci sono Comuni piccoli come Pozzuoli che hanno maturato una perdita potenziale di qualcosa come 18,820

Signor Presidente, vorrei semplicemente riferire della preoccupazione che il Gruppo del Partito Democratico avverte, mio tramite, per le sorti della Scuola italiana di archeologia in Atene.

e quindi ci priveremmo di un avamposto significativo sotto il profilo culturale. Vorrei che il Governo considerasse l’ipotesi, affacciata dall’emendamento a mia firma, di incrementare il fondo di 500.000 euro l’anno per ciascuna delle tre annualita2009, 2010 e 2011. Il collega senatore Francesco Rutelli,

quanto sia valida e significativa la presenza in Grecia di un’istituzione culturale come la Scuola italiana di archeologia in Atene. Vorrei quindi pregare l’onorevole Sottosegretario

interventi sulla fiscalita energetica per finalitasociali e misure per favorire l’insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche. L’emendamento 3.Tab.C.34 prevede l’aumento dei fondi assegnati all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi

di incrementare il finanziamento dell’Autorita garante della concorrenza e del mercato. Lo ripeto ancora una volta in quest’Aula. Questo eun Governo allergico alle regole. Abbiamo un’Autorita garante della concorrenza e del mercato che svolge opera

Concludo, signor Presidente, confidando anche nella saggezza di questo Governo, che non mi pare ne abbia molta. Signor Presidente, tratterosinteticamente le modifiche che proponiamo a quattro tabelle (A.10, A.12, A.15 e A.16) e congiuntamente anche le questioni relative a tre ordini del giorno dei quali sono primo firmatario. La manovra finanziaria in esame dispone non soltanto forti riduzioni delle autorizzazioni di spesa relative alle missioni sicurezza e giustizia, ma, fatto piu grave, non prevede alcuna misura a tutela della sicurezza dei cittadini; in aggiunta non prevede norme volte a promuovere e a sostenere il contrasto al crimine organizzato, anche di natura transnazionale. Nel provvedimento in esame, si rileva che sono del tutto assenti norme volte a contrastare e prevenire fenomeni gravemente pregiudizievoli per lo sviluppo economico del Paese, quali l’infiltrazione delle organizzazioni mafiose nell’economia e nel mercato. 2008 evidente a tutti che, al fine di contrastare la criminalitaorganizzata e contenere i gravi pregiudizi che essa arreca allo sviluppo economico del Paese, nonche´ alla liberta, alla sicurezza e all’incolumitadei cittadini, e necessario dotare le forze dell’ordine, la polizia giudiziaria e la stessa magistratura – in particolare, requirente – di risorse adeguate alle funzioni loro attribuite dalle leggi costituzionali e ordinarie. La tendenza sempre piufrequente del crimine organizzato a strutturarsi in una dimensione transfrontaliera dimostra la necessita di potenziare le attivitadi cooperazione di polizia e di polizia giudiziaria in ambito europeo e, in generale, internazionale, favorendo la condivisione di informazioni e il coordinamento delle indagini, anche avvalendosi dell’istituto delle squadre investigative sovranazionali previste dalla decisione-quadro europea del 2002. Di queste esigenze nella manovra finanziaria non c’e assolutamente traccia. Un’altra questione riguarda piunello specifico

concernente l’azione collettiva risarcitoria. In questa manovra finanziaria sono del tutto assenti norme idonee a promuovere l’efficienza dell’amministrazione della giustizia nonche´ a migliorare lo standard della tutela giurisdizionale dei diritti. E, in aggiunta, non vi e alcuna previsione di misure a tutela dei consumatori o, comunque, delle categorie di cittadini lesi da condotte illecite seriali diffuse, quali la class action, azione collettiva a tutela dei consumatori, introdotta dalla legge finanziaria del 2008, pero` attualmente congelata dal Governo e da questa maggioranza.

L’emendamento che intendo illustrare, il 3.Tab.A.21, riguarda un tema che, a prima vista, sembra locale, ma che, come cercherobrevemente di spiegare, assume anche un connotato nazionale ed internazionale. Si tratta, cioe, dell’attenzione – o, piupropriamente, della disattenzione di questo Governo per le minoranze linguistiche. E[ ]stato ridotto ad una cifra irrisoria il fondo previsto dalla legge n. 482 del 1999 per le minoranze linguistiche storiche, come anche quello per la minoranza italiana in Istria. A queste, si aggiunge la minoranza slovena nella Regione Friuli-Venezia Giulia, che, con questa finanziaria, si vede ridurre notevolmente i fondi per le sue attivita. Vorrei sottolineare che il tema proposto riguarda un territorio che nel secolo scorso e stato protagonista di pagine di storia molto dolorose (che hanno provocato sofferenze e drammi da ambedue le parti), ma che fortunatamente oggi guarda al futuro. Negli ultimi anni si erafforzato il processo di pacificazione, convivenza e integrazione; i rapporti fra la Slovenia e l’Italia hanno fatto un salto di qualita, nella reciproca consapevolezza del ruolo che questi due Paesi possono

Questo territorio multietnico puoessere additato come laboratorio ed esempio di pacifica convivenza ai Paesi in cui l’appartenenza etnica rischia ancora sempre di provocare conflitti. ]necessario, percio, garantire alla comunita slovena la tutela dei diritti sanciti dalla Costituzione, dai trattati e convenzioni internazionali, ultimo dei quali eil Trattato di Lisbona. Con la drastica riduzione dei fondi previsti dalla legge n. 38 del 2001, si mette a repentaglio l’attivita di enti ed associazioni culturali, di ricerca, sportive, sociali ed altre, cioe` tutto quel tessuto sociale che, insieme alla scuola e all’uso della lingua, contribuisce a mantenere viva la minoranza stessa. Si chiede al Governo solamente di applicare la legge n. 38, che senza un’adeguata copertura finanziaria diventa solo un’enunciazione di principi. In sintesi, si chiede di ripristinare il capitolo di riferimento al livello previsto dalla finanziaria 2008.

per recuperare tale posizione. Abbiamo parlato molto di sicurezza scolastica nei giorni scorsi, anche a causa di eventi drammatici; abbiamo proposto di destinare il 20 per cento di quello che viene risparmiato nella

l’intervento di una ventina di giorni fa del presidente del CONI al Senato. In merito al taglio di 95 milioni di euro dello sport per tutti, il sottosegretario Crimi aveva promesso

di rendersi disponibile a prendere in esame nuovamente questi argomenti.

il recepimento di un ordine del giorno che vada incontro al senso piu profondo delle nostre proposte, avremo la chiusura pressoche´ immediata

i 200 milioni di euro tagliati alla cooperazione. Ricordo che e stato il Governo Prodi a riportare a livelli

Sappiamo che l’Africa e in gravissimo ritardo su tutti gli obiettivi cosiddetti del millennio. Quindi, la cooperazione assume realmente un ruolo centrale. Noi ci presentiamo a La Maddalena con un pessimo biglietto da visita. Il presidente Berlusconi ebravissimo come anfitrione dei grandi della terra e sono sicuro che la scenografia e la regia

servire. SERRA (PD). Signor Presidente, il ridotto spazio che mi e` stato concesso mi consente soltanto di sottoscrivere quanto sostenuto da autorevoli esponenti, tra l’altro della maggioranza, in Commissione difesa. In quella sede, tutte le parti politiche hanno denunciato i mortificanti tagli operati al settore. Sottolineo, usando le parole di uno dei senatori della maggioranza,

difesa e della pubblica sicurezza. Sono sulla stessa linea il capo di stato maggiore Camporini e tutti i comandanti delle Forze armate intervenuti in Commissione negli ultimi

Ricordo a titolo di esempio che tra le gravi conseguenze della finanziaria denunciate dai vertici delle Forze armate e stato annoverato anche il rischio della chiusura delle scuole di perfezionamento entro il 2010. L’intero arco costituzionale della polizia e le associazioni della difesa hanno stigmatizzato gli indecorosi tagli, ma l’unica risposta giunta dal Governo estata quella di stanziare 12 milioni

Riteniamo che le nostre Forze armate meritino di piu. Se evero che quest’Aula non e divenuta ormai soltanto un luogo di ratifica delle decisioni assunte dal Governo; se evero che la maggioranza auspica un dialogo ed una collaborazione

su questo punto e che certamente non ci si vuole prendere gioco delle Forze armate; ebbene se tutto cio evero, e il tempo di verificarlo.

sono camere private costituite da imprenditori italiani che svolgono la propria attivitain territorio straniero e si organizzano in questo modo, dandosi una forma istituzionale di collegamento con il proprio Paese di origine. La cifra che viene richiesta e modesta ed ecompresa nel capitolo piu generale delle spese per gli interventi per l’internazionalizzazione. Poiche´ peroieri il sottosegretario Vegas ha ricordato che non sono plausibili modifiche della Tabella C, vorrei almeno che su questo argomento si considerasse la possibilita di un ordine del giorno

(PD). Signor Presidente, onorevoli senatori, intervengo per illustrare l’emendamento 3.Tab.A.35, relativo al ripristino del Fondo per lo sminamento umanitario.

11 dicembre 2008 non possiamo essere distratti nell’affrontare questo problema o non sentirci tutti personalmente coinvolti. Stiamo parlando, infatti, di un’attivitache e assolutamente necessaria per ridurre le sofferenze di quelle popolazioni che, giacolpite dagli effetti tragici delle guerre e delle crisi internazionali, continuano a pagare un tributo pesantissimo in termini di vite umane e di infermita permanenti anche dopo la fine di questi conflitti per anni e anni. La presenza delle mine antiuomo accompagna quasi sempre i conflitti tra gli Stati e le etnie ed euna delle cause di maggiore violenza nei confronti delle popolazioni civili che cercano di recuperare, dopo tanti patimenti, una parvenza di serenita e di normalitadi vita. Vorrei sottolineare altresı il fatto che le vittime piunumerose delle mine sono i bambini, che molto spesso con innocenza e inconsapevolezza si avvicinano a quegli ordigni scambiandoli tragicamente per innocui giocattoli. Alcuni dati per configurare la drammatica dimensione del problema: in Bosnia Erzegovina sono stati posati oltre tre milioni di mine durante la guerra degli anni Novanta del secolo scorso e numerose aree sono tuttora interdette all’utilizzazione ed alla coltivazione per la loro presenza. I confini I confini tra il Kosovo e l’Albania sono in larga misura non percorribili, se non nelle limitate vie che sono state gia bonificate. In Afghanistan – questo el’elemento piu drammatico fino a circa qualche mese fa le vittime giornaliere di questa tragica presenza di mine arrivavano a 70 unitaal giorno.

A mio modo di vedere, ripristinare il Fondo per lo sminamento umanitario e per tutti noi, onorevoli senatori, un dovere morale. Non possiamo sottrarci ad esso per tre semplici ragioni: innanzitutto per la contenuta entitadelle risorse che si vuole inserire in tale tabella, pari ad un milione di euro; per il significato morale che avrebbe il reinserire questi fondi; infine, la piu importante delle ragioni: credo che quest’Aula non possa non concordare con quanto da me rappresentato e si intende chiedere attraverso l’emendamento perche´ ela stessa Aula che in passato ha bandito l’impiego delle mine antiuomo e che pochi mesi fa

Nel corso di un’audizione che si esvolta presso la Commissione affari costituzionali del Senato, il sottosegretario Bonaiuti

non possono far parte della legge finanziaria. Pero`, signor Sottosegretario, non ci potevate impedire di intervenire sul rifinanziamento di leggi precedenti

ignorarli totalmente: chiedono di andare a morire nelle proprie case e credo che ne abbiano tutto il diritto. Nel cratere non einiziata la ricostruzione, altro che modello Molise da contrapporre al modello Umbria e Marche, come si e detto negli anni passati!